abbiamo avuto anche dei lutti e non ho la pretesa di esaurire un elenco che sarebbe più lungo. Voglio comunque ricordare che venerdì 4 agosto è mancato Nicola Conte, papà di Giuseppe Conte, presidente del MoVimento 5 Stelle. A lui e al Gruppo rivolgo le condoglianze a nome del Senato. Il 14 agosto è morto, all'età di novantatré anni, il professor Francesco Alberoni, grande sociologo e scrittore. Il Gruppo Fratelli d'Italia mi ha chiesto di ricordarlo la prossima settimana,

Il 17 agosto, sulle Alpi Giulie, sono mancati due agenti della Guardia di finanza durante un addestramento. sapete, giovedì 31 agosto, a Brandizzo, sulla linea ferroviaria Torino-Milano, cinque operai, Kevin Laganà, Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Giuseppe Saverio Lombardo e Giuseppe Aversa, hanno perso la vita in un drammatico incidente. Per tutti loro, ma anche per le altre sei donne uccise in episodi di femminicidio nel solo mese di agosto, Iris Setti, Maria Costantini, Celine Frei Matzohl, Anna Scala, Vera Schiopu, Francesca Renata Marasco e, ieri, Rossella Nappini, credo credo che sia sentito, da parte di tutto il Senato, rivolgere un pensiero e osservare un minuto di silenzio.

Il sottosegretario Tripodi si è associato, a nome del Governo. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. Comunico che in data 11 agosto 2023 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro delle imprese e del made in Italy*, *dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'interno, dal Ministro del turismo, dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*, *dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro della salute e dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica* Italy Urso Adolfo ed altri Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici che è stato già presentato alla Camera dei deputati lo scorso 10 agosto. Comunico altresì che in data 31 agosto è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze* «Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, recante misure urgenti in materia di finanziamento

un'alta presenza di senatori e di questo vi ringrazio.

L'Assemblea è chiamata ed esaminare il disegno di legge di iniziativa governativa recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Repubblica del Kosovo in materia di cooperazione di polizia, sottoscritto dalle parti L'Accordo oggi al nostro esame risponde all'esigenza di intensificare la cooperazione tra le Forze di polizia dei due Paesi per promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione bilaterale, al fine di prevenire e contrastare la criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme e il terrorismo internazionale. L'Accordo, che si inserisce in un contesto internazionale che richiede una sempre maggiore collaborazione fra i Paesi nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, costituisce lo strumento giuridico per regolamentare la collaborazione operativa e per rafforzare i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati in questa lotta. L'Intesa bilaterale promuove, sviluppa e rafforza la collaborazione di polizia per la prevenzione e il contrasto della criminalità nelle sue forme e del terrorismo, individuando le autorità competenti responsabili della sua attuazione. L'Accordo indica inoltre i principali settori entro i quali la cooperazione di polizia si svilupperà: il contrasto al crimine organizzato transnazionale, i reati contro la vita, l'incolumità personale e l'integrità fisica, la produzione e il traffico illecito di stupefacenti, la tratta di persone e il traffico illecito di migranti, nonché di armi, la criminalità informatica e la pedopornografia *online*, i reati economici e finanziari e il terrorismo. L'intervento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Dreosto. Ne ha facoltà.

sulla cooperazione di polizia si intende evidentemente creare le condizioni per una maggiore cooperazione tra le Forze di polizia dei due Paesi È fondamentale prevenire e contrastare le attività di criminalità organizzata transnazionale in un'area strategica per gli interessi del nostro Paese come quella del Kosovo e dei Balcani in generale. Per queste ragioni, con tale Accordo l'Italia dimostra ancora una volta di voler intensificare le proprie collaborazioni e attività per una maggiore stabilità dei Balcani che importante ricordarlo - fanno parte di quel Mediterraneo allargato che è una priorità imperativa della nostra politica estera e di difesa. L'Accordo è volto non solo al contrasto della criminalità organizzata, ma anche delle attività del terrorismo internazionale che purtroppo è riuscito ad infiltrarsi in Paesi del nostro vicinato. Nonostante un'attenzione centrata sul fronte Est, è necessario non sottovalutare questa costante minaccia che il terrorismo, in particolare di natura jihadista,

che purtroppo in questo periodo è terra di arrivo di migranti provenienti proprio dalla cosiddetta rotta balcanica e che quindi è messo a dura prova dal costante aumento dei flussi migratori che percorrono i Balcani fino ad arrivare ai confini nord-orientali del nostro Paese, raggiungendo poi le Province di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine. Ecco che quindi c'è la possibilità che tra questi migranti vi siano anche criminali, soggetti pericolosi e terroristi internazionali che si infiltrano con lo scopo di arrivare sul suolo italiano ed europeo, intensificando così quella rete criminale ed eversiva che mette a repentaglio la sicurezza del nostro Paese e dei nostri cittadini. Per queste ragioni, ben vengano accordi come quello tra l'Italia e il Kosovo e anche altri Paesi dei Balcani per intensificare le operazioni di polizia *in loco*.

e non possiamo più piegarci alla volontà delle ONG, delle reti di criminali, organizzazioni terroristiche o altri attori statuali ostili, su una tematica così importante ed estremamente sensibile per il nostro Paese.

provvedimento strategicamente importante anche perché va a chiudere un accordo di cooperazione su temi importanti, quale ad esempio il contrasto al crimine in varie sue forme e declinazioni, ampliando

risalente al settembre 2021, dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva sottoscritto dall'Italia e dalla Repubblica di San Marino nel marzo 2008. L'obiettivo sotteso al Protocollo emendativo è quello di rafforzare la cooperazione in materia radiotelevisiva tra le due società concessionarie del servizio pubblico, nell'interesse dello sviluppo culturale, economico e sociale dei due Stati. L'iniziativa risponde, in particolare, all'esigenza di innovare l'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva del 2008 per l'intervenuta necessità di ridefinire l'assetto delle frequenze radiotelevisive, allo scopo di consentire la realizzazione del sistema 5G in Italia. È evidente a tutti che si tratta di un settore in continua evoluzione tecnologica, per cui un accordo del 2008 è evidentemente da considerarsi Il Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva, oltre a estendere la vigenza dell'Accordo prolungandola al 2026, prevede in particolare alcuni impegni rilevanti per i due Paesi, come la conferma della rinuncia da parte di San Marino all'utilizzo di alcuni dei propri canali televisivi e la rinuncia all'uso di quelli digitali radiofonici, a fronte, da parte italiana, dell'impegno alla ritrasmissione sull'intero territorio italiano del segnale televisivo della San Marino RTV, con contestuale riconoscimento di un incremento del contributo economico annuale con decorrenza dall'anno 2021. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

la ratifica del Protocollo emendativo che a breve ci accingeremo a votare ha lo scopo di rafforzare la cooperazione in materia radiotelevisiva fra le due società concessionarie del servizio pubblico, aggiornando l'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva del 2008 per intervenuta necessità di modificare l'assetto delle frequenze radiotelevisive allo scopo di consentire la realizzazione del sistema 5G. In tale contesto, l'analisi tecnico-normativa sottolinea che il canale 51, il cui uso su parte del territorio italiano è stato riconosciuto a San Marino dall'Accordo attuale, dovrà essere dismesso per consentire al nostro Paese di dedicare le relative frequenze al nuovo sistema 5G. Il Protocollo impegna quindi l'Italia a facilitare la conclusione di un accordo tra la San Marino RTV e un operatore nazionale italiano al fine di assicurare il trasporto di un programma di San Marino RTV su una rete che

culturale tra i due enti concessionari del servizio pubblico RAI e la San Marino RTV. Il Protocollo, oltre a estendere al 2026 la vigenza dell'Accordo, prevede anche alcuni impegni rilevanti per i due Paesi, come la conferma della rinuncia da parte di San Marino all'utilizzo di alcuni canali televisivi e ai canali digitali radiofonici, a fronte dell'impegno italiano alla ritrasmissione sull'intero territorio italiano del segnale televisivo della San Marino RTV, con contestuale riconoscimento di un incremento del contributo economico annuale. Aggiungo che il provvedimento in oggetto nasce da un'iniziativa legislativa assunta dalla Lega attraverso una proposta di legge presentata dall'onorevole Formentini, che ringrazio, avente ad oggetto lo stesso contenuto, che venne approvata la scorsa legislatura, nel corso della seduta del 22 marzo 2022, dalla Commissione

Presidente, Governo, colleghi senatori, oggi trattiamo la ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino. Il disegno di legge di ratifica è composto da quattro articoli. L'articolo 1, denominato «Autorizzazione alla ratifica», prevede la dismissione del canale 51 per consentire al nostro Paese di dedicare le relative frequenze al nuovo sistema 5G il relativo impegno del nostro Paese a facilitare le conclusioni di un accordo tra lo Stato di San Marino e l'operatore nazionale italiano, al fine di assicurare il trasporto di un programma di San Marino RTV su una rete che fornisca la copertura di ambito nazionale nel territorio italiano. L'articolo 2 prevede l'ordine di esecuzione del protocollo stesso. L'articolo 3 stabilisce il contributo economico che lo Stato italiano si impegna a versare annualmente allo Stato sammarinese:

Di contro, lo Stato di San Marino rinuncia all'utilizzo di alcuni canali televisivi e canali digitali radiofonici. L'Italia quindi si impegna alla ritrasmissione sull'intero territorio italiano del segnale televisivo della RTV San

del disegno di legge n. 684. La relatrice facente funzioni, senatrice Craxi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge di iniziativa parlamentare recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Costa Rica sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, sottoscritto nel maggio 2016. L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica si propone di fornire un quadro giuridico di riferimento per lo sviluppo dei rapporti tra l'Italia e la Costa Rica in questi settori, al fine di rinsaldare e intensificare i legami di amicizia già esistenti e migliorare ulteriormente il quadro delle relazioni bilaterali. L'intesa bilaterale esplicita innanzitutto l'impegno delle parti a promuovere la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico, a migliorare la conoscenza, la diffusione delle rispettive lingue e culture e a favorire la collaborazione tra rispettive istituzioni accademiche, amministrazioni archivistiche, biblioteche e musei. Le parti possono inoltre chiedere la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento dei programmi promossi nell'ambito delle forme di cooperazione individuate dall'Accordo e delle attività di istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi, il rafforzamento della collaborazione nel campo dell'istruzione mediante lo scambio di esperti, di informazioni e documentazioni sulle rispettive legislazioni, anche al fine di sottoscrivere accordi per il riconoscimento e l'equiparazione dei titoli universitari e l'offerta di borse di studio. L'Accordo impegna inoltre le parti alla collaborazione reciproca nel settore editoriale, nella musica, nel cinema, nelle arti visive e nell'ambito radiotelevisivo, nonché a impedire e reprimere l'importazione, l'esportazione e il traffico illegale di opere d'arte. Ulteriori ambiti di collaborazione e di scambio di esperienze interessano i settori dello sport e della gioventù, dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché delle pari opportunità e della tutela delle minoranze. La promozione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, in particolare nei campi delle tecnologie, dell'informazione e della multimedialità applicata all'informatica, alla biomedica e ai beni culturali, consentirà la stipula di specifici accordi tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche nei due Paesi. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

l'Accordo istituisce un quadro giuridico di riferimento per lo sviluppo dei rapporti tra l'Italia e la Costa Rica nei settori della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, al fine di rinsaldare ed intensificare i legami già esistenti e di migliorare ulteriormente il quadro delle relazioni bilaterali. Anche su questo vi è la dimostrazione cristallina di come l'attività diplomatica italiana agisca a 360 gradi e sia rivolta non solo al nostro vicinato, ma anche ad altre aree chiave per la difesa dei territori nazionali, interessati come l'America centrale. I settori in cui eccelliamo, come quello culturale, scientifico e tecnologico, ci permettono di continuare un'azione di accrescimento del nostro *soft power* e di mantenere buone relazioni bilaterali con Paesi quali la Costa Rica.

Signor Presidente, questo disegno di legge a mia prima firma ha lo scopo di ratificare l'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica firmato a Roma il 27 maggio 2016 fra il Governo italiano e il Governo della Costa Rica. Le relazioni bilaterali fra questi due Paesi sono solide, cordiali e improntate a un fiducioso rapporto di grande amicizia e collaborazione. ottimo andamento è confermato anche dalla piena collaborazione soprattutto nei fori multilaterali, con numerosi casi di sostegno reciproco alle rispettive candidature internazionali. Basti ricordare l'appoggio della Costa Rica alla candidatura italiana al consiglio di sicurezza dell'ONU, cinque anni fa. Inoltre, tali relazioni sono favorite dai solidi rapporti commerciali fra i due Paesi. La Costa Rica è difatti il quarto più importante *partner* dell'Italia in Centro America, dopo Messico, Panama e Cuba, con un interscambio globale che solo nel 2015 2015 (l'anno prima della firma) ha raggiunto la cifra *record* di 379,5 milioni di euro. L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica si inserisce quindi nel contesto di un rilancio delle relazioni bilaterali dell'Italia con uno dei *partner* tradizionali dell'America centrale, un Paese che si caratterizza per la stabilità politica e gli indici di sviluppo tra i più elevati di quell'area. Non è mai stato firmato prima uno specifico accordo nel settore, perché esisteva un accordo quadro tra Italia e Costa Rica, firmato il 24 ottobre 1983, che riguardava principalmente la cooperazione economica, finanziaria, sociale e culturale. si compone di 21 articoli. Fra essi, alcuni sono di fondamentale importanza per rinsaldare ancor di più i rapporti fra i due Paesi. Gli articoli da 1 a 3 definiscono l'impegno delle parti a promuovere la cooperazione nei settori indicati, a migliorare la conoscenza e la diffusione delle rispettive lingue e culture e a favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche, amministrazioni archivistiche, L'articolo 4 prevede la possibilità, per le parti, di chiedere la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento dei programmi promossi nell'ambito delle forme di cooperazione individuate dall'Accordo. L'articolo 5 disciplina la possibilità reciproca di istituire attività di istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi. Gli articoli da 6 a 8 hanno lo scopo di rafforzare la collaborazione nel campo dell'istruzione, mediante lo scambio di esperti, di informazioni e di documentazione, anche al fine di sottoscrivere accordi per il riconoscimento e l'equiparazione dei titoli universitari e l'offerta di borse di studio. L'articolo 19 affida a una commissione mista lo sviluppo della cooperazione culturale, la redazione di programmi esecutivi pluriennali e la valutazione dello stato di attuazione L'articolo 20 riguarda l'applicazione e l'interpretazione del testo. Infine, l'articolo 21 disciplina la durata, che è illimitata, e le modalità di modifica dell'Accordo. Presidente, la Costa Rica è uno dei Paesi che ho l'onore di rappresentare in Parlamento, perché è della mia ripartizione, della mia circoscrizione elettorale.

che ha dato un sostanziale contributo allo sviluppo del Paese. Nei miei contatti diretti con la collettività italiana in Costa Rica ho appunto potuto riscontrare personalmente quanto sia auspicata la ratifica di questo Accordo, non soltanto dagli oltre 6.000 cittadini italiani che vivono in quel Paese, ma anche per i costaricani che vivono in Italia e per tutte le istituzioni culturali e scientifiche, dalle università agli istituti di ricerca medica e scientifica.

la Repubblica del Costa Rica, che, com'è stato giustamente detto in alcuni degli interventi precedenti, è una delle democrazie più stabili del Centro America e addirittura complessivamente dell'America Latina, coinvolge Italia e Costa Rica in una innumerevole serie di settori (culturali, scientifici, accademici, museali e archivistici).

Penso all'articolo che prevede la possibilità di istituire scuole italiane in Costa Rica, che credo vada nella giusta direzione per dare sponda e margine alla diffusione della nostra cultura. Pertanto, è evidente che non possiamo che guardare con favore a questo tipo di iniziativa. Le altre innumerevoli materie materie enunciate e declinate nei 21 articoli di questo Accordo sono già state citate dagli interventi precedenti, quindi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

fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021*** *(Approvato dalla